La seduta è aperta

colleghi, comunico di aver ricevuto la seguente lettera dal Presidente del Consiglio dei ministri: «Roma, 26 febbraio 2007 Onorevole Presidente, La informo che il Presidente della Repubblica ha respinto le dimissioni da me rassegnate in data 21 febbraio scorso

la seduta sarà sospesa per consentire all'onorevole Prodi di recarsi alla Camera dei deputati per la consegna del testo del proprio intervento. La seduta riprenderà alle ore 18,30 per l'avvio della discussione generale che proseguirà questa sera fino alle ore 20,30, quindi domani, dalle ore 9,30 alle ore 14 e dalle ore 16 alle ore 18. Dalle ore 18 di domani avranno luogo la replica del Presidente del Consiglio dei ministri e le dichiarazioni di voto, con trasmissione diretta televisiva. Si procederà, quindi, alla votazione nominale con appello. I tempi per la discussione generale e per le dichiarazioni di voto sono già stati comunicati ai Gruppi. Resta fermo per giovedì mattina l'esame del decreto-legge sulle competizioni calcistiche, ove concluso dalle Commissioni riunite. Si aggiunge, poi, per la prossima settimana il decreto-legge sull'attuazione di obblighi comunitari ed internazionali.

Signor Presidente del Senato, onorevoli senatrici e onorevoli senatori, l'Esecutivo da me presieduto è stato nei giorni scorsi messo in minoranza in una votazione che aveva per oggetto un capitolo fondamentale dell'azione di Governo e della vita del Paese: la politica estera e di sicurezza. Già prima del voto, nella maggioranza si erano, tuttavia, manifestate tensioni, con un'accentuata litigiosità tra le diverse componenti. Per questo motivo non ho, sin dall'inizio, nascosto la natura politica di questa crisi e ho immediatamente presentato le dimissioni al Capo dello Stato. Al termine delle approfondite consultazioni e dopo aver ascoltato tutte le formazioni politiche presenti in Parlamento, il presidente Napolitano ha respinto le dimissioni e ha rinviato il Governo alle Camere, anche in virtù del chiarimento politico avvenuto nel frattempo tra le componenti della maggioranza. Sono qui oggi, dunque, per chiedere il rinnovo della fiducia, per restituire immediata e piena normalità all'attività parlamentare, per riprendere con determinazione e slancio ancora maggiori l'azione di Governo. Signor Presidente, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, ho affermato che questa è una crisi politica. Ciò richiede che il Governo e la maggioranza che lo sostiene ne traggano fino in fondo gli insegnamenti conseguenti: insegnamenti di metodo e gli insegnamenti di merito. La prima lezione che dobbiamo trarre è che questa crisi si colloca all'interno della lunga ed incompiuta transizione del sistema istituzionale e politico del Paese avviata nei primi anni Novanta. Ebbene, uno dei nodi principali di questa transizione è rappresentato dall'attuale legge elettorale. Per questo motivo, rispondendo con convinzione all'invito del Presidente della Repubblica, ribadiamo l'impegno con il quale ci siamo presentati alle elezioni e consideriamo come nostro dovere quello di operare per una pronta riforma del sistema elettorale. Su questo argomento, tuttavia, mi soffermerò a conclusione del mio intervento. Ora vorrei parlarvi di quelli che d'ora in avanti dovranno essere il metodo e il merito dell'azione del Governo e della maggioranza. Le forze che sostengono il Governo hanno ispirazioni culturali differenti, ma tutte sono accomunate da un obiettivo di riforma e di profondo rinnovamento del Paese. Questo obiettivo non potrà essere perseguito se non si avrà come unico punto di riferimento l'interesse generale della comune azione di Governo. All'interno dell'Esecutivo e della maggioranza sono e saranno garantiti spazi e occasioni per un confronto aperto delle posizioni e delle proposte ma, una volta giunti ad una sintesi e ad un'intesa, essa sarà da tutti seguita e rispettata. Lo scorso 21 febbraio è sulla politica estera che si è determinata la crisi. È giusto pertanto che sia proprio da qui, dalla politica estera, che noi, Governo e maggioranza, riprendiamo il nostro cammino, ricordando quanto abbiamo fatto fin ad ora e annunciando con chiarezza cosa intendiamo fare nel futuro. Il 12 dicembre del 2003, in una situazione di forte polarizzazione del rapporto tra Europa e Stati Uniti, il Consiglio europeo adottò, per la prima volta nella sua storia, una strategia di sicurezza comune. Il concetto chiave su cui si basava questa strategia era il multilateralismo: nessun Paese europeo, preso singolarmente è, infatti, in grado di affrontare e risolvere problemi di portata mondiale. Nel definire la politica estera e di sicurezza del nostro Governo, fu quello il concetto essenziale al quale noi ci siamo sempre rifatti. Abbiamo perciò collocato l'Italia al centro dell'Europa, costruendo un rapporto stretto con Germania, Francia e Spagna, senza per questo allentare le relazioni con il Regno Unito. E noi guardiamo all'Alleanza Atlantica e agli Stati Uniti come complemento naturale della scelta europea, in coerenza con la politica estera e di sicurezza che ha guidato tutta la nostra storia repubblicana. Coerenti con questo quadro, ribadiamo gli impegni che da questi rapporti ci derivano con gli Stati Uniti e, partendo da tali principi, abbiamo sviluppato la nostra azione nelle aree a noi più immediatamente vicine. Nei Balcani abbiamo perseguito un'azione volta a favorire la definitiva stabilizzazione della regione, avendo in mente la prospettiva di adesione di tutti questi Paesi all'Unione Europea. Parlando del Medio Oriente, non posso non ricordare la decisione di portare a compimento la missione in Iraq con il rientro delle nostre truppe; rientro avvenuto in modo concordato con le autorità irachene, senza creare vuoti di sicurezza. In Medio Oriente abbiamo sviluppato una politica di attenzione verso tutti gli attori della regione, convinti che il miglior modo per aiutare la pace e la stabilità della regione stessa non è quello di scegliere una parte a scapito dell'altra, ma, al contrario, quello di sforzarci di capire le ragioni degli uni e degli altri. Questo è l'unico metodo in grado di far progredire il cammino della pace. Non si tratta di retorica, ma di un metodo coerente di lavoro: la decisione di assumere una posizione di guida nell'invio di una missione di *peace-keepers* in Libano sotto l'egida delle Nazioni Unite ne è un'applicazione concreta. Considero questa decisione uno dei momenti più significativi dell'azione di politica estera del nostro Governo. Essa è stata sviluppata nell'ambito delle Nazioni Unite, d'intesa con i nostri *partners* europei, con il pieno sostegno di Washington, Mosca, Pechino e di molti Stati musulmani e con l'appoggio convinto delle parti, Libano e Israele, così come degli altri attori regionali. Abbiamo dimostrato che siamo capaci di assumerci responsabilità importanti e di svolgere un'azione di guida senza mai abbandonare l'approccio multilaterale. Ma abbiamo anche dimostrato che questo Governo è pronto a utilizzare le proprie truppe quando si tratta di porle con generosità al servizio della pace e della stabilità. Guardando ora al futuro - e sempre rimanendo nella regione mediorientale - voglio confermare che continueremo ogni sforzo per avvicinare le posizioni di israeliani e palestinesi e rendere finalmente possibile la prospettiva di due Stati e due popoli che possano vivere in pace e sicurezza l'un accanto all'altro. Siamo ugualmente impegnati a tenere aperto un canale di dialogo con l'Iran. Se è vero che le scelte di Teheran hanno creato una situazione di forte contrapposizione con la comunità internazionale, è anche vero che occorre fare tutto il possibile per evitare il precipitare della crisi verso una soluzione militare. Non voglio sfuggire alla questione della nostra presenza in Afghanistan. Sono ben cosciente che si tratta di un tema su cui esistono sensibilità diverse e sono convinto che la presenza militare non possa rappresentare, da sola, la soluzione ai problemi della Regione. Il Governo ha sostenuto con convinzione - e continuerà a farlo che solo un'azione politica che coinvolga tutta la comunità internazionale (e in particolare i Paesi confinanti) potrà garantire la stabilità dell'area. È questo il senso della conferenza per la pace in Afghanistan, conferenza che stiamo proponendo da tempo. Una proposta che, dopo la fatica iniziale, sta raccogliendo consensi crescenti, a partire da quello espressomi personalmente dal presidente Karzai. La nostra presenza in Afghanistan ha l'obiettivo di aiutare e sostenere il processo di consolidamento delle giovani istituzioni democratiche del Paese. I nostri soldati in Afghanistan - come in tutte le nostre missioni - sono portatori di una cultura di dialogo e di aiuto, non di confronto o di scontro. A loro va un'ammirazione che so essere condivisa da tutte le forze politiche di questo Parlamento. si parla di pace e stabilità, occorre parlare anche di solidarietà e cooperazione e io penso in particolar modo al Continente africano. Nei mesi scorsi abbiamo già fornito un concreto segnale di sostegno all'Africa raddoppiando i fondi del nostro aiuto pubblico allo sviluppo, portandoli a 700 milioni di euro per il 2007. Abbiamo anche voluto far fronte agli impegni assunti internazionalmente, versando al Fondo globale per la lotta all'AIDS, alla tubercolosi e alla malaria, i 260 milioni di euro che rappresentano la nostra quota per gli anni 2005, 2006 e 2007. Anche sul piano più propriamente politico abbiamo dato un segnale preciso con la mia partecipazione, unico Capo di Governo dell'Unione Europea, al vertice dell'Unione Africana di Addis Abeba. Il nostro obiettivo è stato e sarà duplice: da un lato, aiutare a costruire un partenariato euro-africano basato sullo sviluppo, sulla giustizia e sui diritti; dall'altro, aiutare la risoluzione di crisi come quella del Darfur e quella del Corno d'Africa, così vicina a noi. Con i nostri *partner* mondiali ci stiamo impegnando per favorire il ritorno a un vero sistema multilaterale per poter affrontare insieme le grandi sfide dell'umanità: i cambiamenti climatici, la lotta alle pandemie, la gestione dei flussi migratori. Abbiamo ingaggiato, in questi mesi, una significativa battaglia contro la pena di morte. Con la nostra proposta di moratoria all'Assemblea generale delle Nazioni Unite siamo diventati capofila di una grande battaglia di civiltà; battaglia di lungo periodo, che ha bisogno di tutte le energie disponibili: politiche, culturali e religiose. Il nostro impegno in campo internazionale non sarebbe completo se non menzionassimo l'impegno per sostenere e valorizzare il patrimonio rappresentato dalle comunità italiane nel mondo, un patrimonio che pochi altri Paesi possono vantare, ma che noi tutti, nei decenni scorsi, abbiamo largamente trascurato. La presenza, per la prima volta in questo Parlamento, di senatori e deputati eletti all'estero è il segno felice di un'inversione di tendenza che dobbiamo onorare e che noi onoreremo. Questi sono alcuni dei punti cardine della nostra politica estera e di sicurezza che fa perno intorno all'articolo 11 della della Costituzione, che si basa sulla profonda convinzione che il quadro multilaterale è il solo che permette di far progredire i processi di riconciliazione nei Paesi in conflitto, di difendere i diritti umani, di abbattere il muro della povertà. Io penso che una politica matura della pace vada giudicata nel suo disegno complessivo e non solo sulle singole scelte. Non chiedo sconti, chiedo solo che si ragioni sulle soluzioni concrete, realistiche e possibili. Questa è la via della pace, questa è la fatica della pace. E ora, è giunto per me il tempo di illustrare gli altri temi e gli altri campi dell'azione di Governo: l'economia, l'ambiente, il Mezzogiorno, l'energia e la ricerca, con una breve premessa e una precisazione. Le parole che oggi vi rivolgo debbono essere lette in continuità con quelle da me qui pronunciate nelle considerazioni programmatiche dello scorso mese di maggio. Il programma di Governo è e rimane il punto di riferimento della nostra azione. Ma, proprio perché esso è già un punto di riferimento condiviso, oggi non ne ripercorrerò, uno per uno, i capitoli. Vi chiedo, pertanto - e lo chiedo, prima che ad ogni altro, ai parlamentari della maggioranza e agli stessi membri del Governo - di non giudicare il mio discorso per quello che esso non contiene. Oggi mi concentrerò su alcune sfide che il corso degli avvenimenti e le novità politiche degli ultimi giorni ci stanno ponendo davanti con maggiore urgenza e intensità. Tra l'ottobre e il dicembre dello scorso anno - e qui vengo all'economia - il Paese ha accelerato il proprio ritmo di crescita, tanto da portare il tasso di sviluppo sul totale dei dodici mesi al 2

e per quest'anno speriamo e, ragionevolmente, pensiamo di fare ancora meglio. So troppo bene che la nostra ritrovata capacità di crescere dipende anche dal positivo andamento dell'economia mondiale ed europea e sono anche consapevole che non tutto il merito dei buoni risultati può essere attribuito al nostro Governo *(Ilarità Colleghi, ho 62 iscritti a parlare e 13 per dichiarazione di voto. Ce n'è di tempo per rispondere!

Tuttavia, posso con tranquilla coscienza affermare che l'azione del Governo ha positivamente stimolato la crescita economica mettendo, contestualmente, sotto controllo i conti pubblici e mantenendo così gli impegni presi con l'Unione Europea. Abbiamo avviato un riordino del sistema delle autorità indipendenti creando, tra l'altro, una speciale Commissione bicamerale per le liberalizzazioni e l'apertura dei mercati. Abbiamo aperto alla concorrenza e liberato da regole e vincoli ormai superati molti settori. Ogni azione in questo campo è stata orientata a favorire il cittadino consumatore che già ne ha tratto concreti benefici, e noi proseguiremo su questa strada.

All'Unione Europea, che per bocca del commissario agli affari economici Almunia ha riconosciuto che l'Italia "sta andando nella giusta direzione", assicuriamo che continueremo a fare la nostra parte con serietà e impegno. Il Governo, ma direi tutta la classe politica del Paese, ha oggi una grande responsabilità, quella di non vanificare gli importanti risultati fin qui conseguiti. Dobbiamo consolidare la crescita economica e dobbiamo completare il processo di risanamento della finanza pubblica. Abbiamo, infatti, un debito pubblico ben superiore alla ricchezza che il Paese è in grado di produrre in un anno. Per ottenere tali obiettivi abbiamo bisogno di coinvolgere tutte le fasce di popolazione, aumentando la loro partecipazione alla vita attiva e la loro produttività. Abbiamo per questo bisogno del contributo di tutti, secondo la specificità di ciascun territorio. Ciò mi porta a toccare in particolare il tema del Mezzogiorno perché lo sviluppo del Mezzogiorno mantiene un'importanza centrale nel programma del Governo. Oltre alle misure previste dalla finanziaria - e penso in particolare alle risorse certe per le infrastrutture stradali e portuali - abbiamo adottato il Quadro strategico nazionale per il 2007-2013 per l'allocazione dei Fondi comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate. Si tratta, complessivamente, di 123 miliardi di euro. È un volume di risorse straordinario, di cui dovremo fare buon uso e dovremo rendere conto. Il Governo è comunque consapevole che una politica per il Mezzogiorno deve puntare in primo luogo e con forza sulla creazione di condizioni di sicurezza per le persone, per gli investimenti e per le imprese. Senza sicurezza non vi sarà sviluppo, così come in passato non vi è stato sviluppo nelle aree in cui l'illegalità ha agito da padrona. I profondi cambiamenti climatici in atto ci impongono l'assunzione di chiari impegni a difesa dell'ambiente, in particolare delle energie rinnovabili e di lotta all'inquinamento. Il pacchetto energia, recentemente approvato dal Governo, va in questa direzione. In particolare, esso punta alla riqualificazione degli edifici, all'aumento dell'efficienza dei consumi industriali, alla mobilità sostenibile. Ma noi non ci possiamo e non ci dobbiamo accontentare. Dobbiamo fare di più e assumere la questione ambientale come una questione centrale dell'Italia e una grande opportunità per la qualità della vita, ma anche per la competitività e per l'innovazione. Penso, ad esempio, ad un grande sforzo di ricerca per le energie rinnovabili di ultima generazione: una nuova energia pulita, abbondante e nelle mani dei cittadini. Dentro a un più profondo impegno nella ricerca e nell'innovazione intendiamo lanciare un progetto di investimento nell'energia solare di ultima generazione. In questo campo, come nel campo della medicina dove in alcuni settori, come la medicina rigenerativa, abbiamo la concreta possibilità di recuperare il terreno da noi in passato perduto. Una politica che limiti il ricorso ad energie altamente inquinanti esige però nel breve e nel medio termine di poter fare uso di fonti più pulite e già oggi largamente disponibili, come il gas naturale. Coinvolgendo e responsabilizzando le autorità locali, procederemo per dotare l'Italia di strutture adeguate allo scopo, dalle reti europee ai terminali. Tra gli impegni internazionali che l'Italia intende rispettare vi è anche il completamento, nei tempi prestabiliti, delle tratte di competenza italiana della rete transeuropea di trasporto. L'Italia farà la sua parte perché le tratte transfrontaliere da Torino a Lione, da Verona a Monaco di Baviera e da Trieste a Divaccia vengano cantierate e concluse nei tempi più rapidi possibili. *(Applausi del senatore Asciutti).* Nello stesso tempo, dovranno essere completate anche le tratte interne, oltre che avviate le "autostrade del mare" da cui dipenderà lo sviluppo del Mezzogiorno. È un impegno assunto in sede europea, e che porteremo avanti con il metodo che noi abbiamo scelto, di un dialogo continuo e aperto con le comunità interessate. I giovani, le donne, gli anziani e le famiglie sono i soggetti e le componenti della nostra società verso cui concentrare uno sforzo straordinario. In particolare, l'Italia registra ancora un grave ritardo per quanto riguarda il ruolo delle donne. Il Governo ha cominciato a lavorare per porre rimedio a queste situazioni, ma molto dovrà e sarà fatto anche in futuro. Affronteremo inoltre, con numerosi strumenti, il tema delle pensioni più basse e delle carriere professionali dei nostri giovani, in particolare di coloro che vivono il dramma della precarietà, perché l'Italia deve sentire il dovere morale di concedere ai propri figli l'opportunità di costruirsi il futuro in dignità e serenità e di impedire che un'intera generazione di giovani affronti la vita senza certezze. A questo ci dedicheremo nell'ambito del riordino del sistema previdenziale e delle politiche del lavoro. Noi ci sentiamo fortemente impegnati per garantire la tenuta finanziaria del sistema, ma, allo scopo di assicurare una maggiore efficienza e ottenere gli indispensabili risparmi, non indietreggeremo di fronte a scelte e a interventi di riorganizzazione anche non facili, come l'unificazione degli enti previdenziali e assistenziali. Come dicevo in precedenza, la crescita va incentivata ulteriormente, ma anche governata con la costante ricerca di maggiore equità e coesione sociale, al centro della quale continuiamo a ritenere debba stare la famiglia. Il rilancio economico, sostenuto da un solido risanamento dei conti pubblici e da una seria, determinata e costante lotta all'evasione fiscale è l'unica condizione per potere ridurre progressivamente il carico fiscale che grava sulle famiglie italiane. Proseguendo poi sulla strada intrapresa negli scorsi mesi, le politiche del Governo si concentreranno con ancora maggiore attenzione sul sostegno alle famiglie e sulla creazione di condizioni e servizi migliori a favore della natalità. L'area delle famiglie interessate all'aumento delle erogazioni monetarie sarà allargata, con l'obiettivo di una loro estensione universale. Inoltre, aumenteremo in modo significativo il numero degli asili nido. La casa ha assunto ancor più che nel passato un peso centrale nel determinare le condizioni di vita reali delle famiglie e richiede un ampio sforzo per affrontare sia le emergenze abitative in senso stretto che le difficoltà nel mercato degli affitti. Rilanceremo perciò l'offerta di edilizia residenziale pubblica, assieme a misure per allargare il mercato privato degli affitti, in particolare con una revisione degli incentivi fiscali. Il Governo inoltre proporrà una modifica del calcolo dell'ICI sulla prima casa, modifica che consentirà significative riduzioni in funzione del numero di componenti in funzione del numero di componenti del nucleo familiare. A tutti questi temi, come a quelli che toccano, più in generale, la questione della crescita o della riforma e del rilancio della pubblica amministrazione, ci dedicheremo utilizzando gli strumenti della concertazione. Non per un fatto formale o di semplice ricerca del consenso. "Concertare" significa in primo luogo saper ascoltare e saper comprendere le ragioni di coloro che operano nella società. Nelle prossime settimane daremo perciò il via a questo percorso, che sarà dedicato ai temi della competitività, della produttività e della crescita compatibile del nostro sistema economico. Nella sua storia, e particolarmente in quella più recente, l'Italia ha dato le prove migliori e più alte quando ha saputo mettere in atto un'azione comune e concordata. E' stato così negli anni della ricostruzione. E' stato così negli anni della lotta al terrorismo. E' stato così nello sforzo per entrare nell'Europa dell'euro. Oggi, pur nel legittimo confronto tra le forze politiche, l'Italia ha bisogno di ritrovare quel medesimo spirito di coesione. Le forze dell'ordine sono state, nei mesi scorsi, impegnate, con dedizione e con risultati straordinari, nel contrasto e nella prevenzione del terrorismo. Mentre, interpretando il pensiero di tutti voi, esprimo la solidarietà a coloro che sono stati oggetto di minacce, rinnovo la riconoscenza a tutte le donne e gli uomini che lavorano per proteggerci. *(Applausi

Solo mostrandoci uniti, potremo sconfiggere in modo definitivo il terrorismo. Ugualmente, solo unendo i nostri sforzi e operando insieme potremo consolidare la ripresa in atto e rendere la nostra società più prospera, più equa e, forse, più serena. Voglio riprendere ora il tema della riforma elettorale. È un compito che certamente trascende l'orizzonte, forzatamente di parte, della maggioranza e del Governo, e che coinvolge la scrittura di regole fondamentali su cui l'intero sistema politico deve potersi riconoscere. Il riassetto complessivo dell'ordinamento deve coinvolgere tutte le parti politiche ed avere nel Parlamento la sua prima e principale sede. È importante che questo avvenga in una prospettiva di aggiornamento complessivo del nostro sistema costituzionale e di definitiva conclusione della troppo lunga transizione italiana. Un impegno, questo, che il presidente Napolitano ha indicato a tutto il Parlamento. È vitale, infatti, avere un sistema istituzionale capace di garantire un'effettiva stabilità dell'azione di Governo, di assicurare un ruolo forte ed incisivo all'opposizione e di rispettare il diritto degli elettori di poter chiedere conto dei risultati conseguiti e delle politiche attuate. Occorre finalmente portare a un equilibrio virtuoso il rapporto fra lo Stato, le Regioni e le altre articolazioni territoriali che esprimono la ricchezza di un Paese pieno di potenzialità e di capacità. Questo, eventualmente, anche attraverso una modifica della composizione stessa del Parlamento. Abbiamo bisogno di una Repubblica governante e governabile che assegni allo Stato e al Governo centrale il compito di garantire l'interesse generale, ma capace di coinvolgere i livelli territoriali nell'assunzione delle decisioni che li riguardano e delle quali essi debbono rispondere ai loro cittadini. Abbiamo bisogno di mettere finalmente a punto un sistema di federalismo fiscale che, in un quadro di equità e di coesione nazionale e di valorizzazione dei territori, assegni ai livelli regionali e locali la necessaria autonomia finanziaria e le conseguenti responsabilità nella gestione delle risorse. È in questo quadro che il Governo si impegna a dare rapida attuazione alla parte del programma che riguarda le minoranze linguistiche e le autonomie speciali.

dare al nostro ordinamento repubblicano un assetto coerente con i grandi valori della Costituzione, ma anche con le sfide del nostro tempo. Spetta al Parlamento stabilire con quali modalità, anche organizzative, svolgere questo lavoro. Deciderà il Parlamento se, a questo fine, potrà essere utile individuare al suo interno un luogo in grado di elaborare, come è necessario, un disegno complessivo e coerente. CASTELLI *(LNP)*. Facciamo Il Governo, da parte sua, farà ogni sforzo per accompagnare il Parlamento in una riflessione che dovrà svolgersi in tempi rapidi. Non tocca a me dare indicazioni in merito. Il ministro Chiti ha iniziato a lavorare su questo; continueremo a farlo, sempre consapevoli del rispetto dovuto al Parlamento e della necessità di cercare e trovare su questi temi il più ampio consenso possibile. Noi non abbiamo pregiudiziali se non una: la nuova legge elettorale dovrà essere il frutto di un'ampia convergenza. Le leggi elettorali, come le modifiche alla Costituzione, non dovranno mai più essere decise dalla sola maggioranza. Credo però che alcuni principi possano essere da tutti condivisi. Noi vogliamo una legge che garantisca ai cittadini di poter scegliere non solo un partito, ma anche un programma, una coalizione, una proposta di Governo, un Primo ministro. Il dibattito su questi nodi dura ormai da alcuni decenni. Esso è riuscito persino a trapassare dalla prima alla seconda fase della nostra esperienza repubblicana, senza mai giungere ad una conclusione adeguata alle esigenze del Paese. L'ambizione che possiamo coltivare è che questa legislatura porti finalmente a termine questa lunga, infinita transizione. Al Parlamento e al Governo che saranno capaci di raggiungere questo risultato, il Paese assicurerà riconoscenza e gratitudine. Il mio auspicio è che quel Parlamento sia questo Parlamento. Ed è su tali propositi e su questo programma, onorevoli senatrici e onorevoli senatori, che chiedo, a nome del Governo, la vostra fiducia. Grazie. Grazie, signor Presidente del Consiglio. Sospendo la seduta, fino alle ore 18,30, per consentire all'onorevole Prodi di recarsi alla Camera dei deputati. *(La

non è possibile chiedere una fiducia che si ha, a meno che il Governo la chieda sulla votazione di un articolo o di un emendamento, ed è legittimissimo che ponga la questione di fiducia su questo. Essendovi in questo momento un unico documento sottoposto al vaglio dell'Assemblea, che è la mia proposta di risoluzione, non risultandone altri, ho motivi di ritenere che, quindi, la fiducia sia stata posta sull'unico documento

così, magari sono pessimista, invece il Presidente del Consiglio la pensa diversamente), dovrei pensare che la fiducia sia stata posta sul diniego alla mia proposta. Altre interpretazioni, Presidente, non ce ne sono e il Resoconto stenografico ha riportato tutto ciò che è stato detto. Senatore Calderoli, ammiro la sua creatività interpretativa regolamentare perché effettivamente c'è del genio. No, qui la No, qui la situazione mi pare sia molto più semplice; è corretto il suo richiamo all'articolo 105 del Regolamento. Come lei ben sa, il Governo è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica dopo le dimissioni rese dal Presidente del Consiglio. Non rileggerò il comunicato del Presidente della Repubblica che è già stato letto dal presidente Marini all'inizio della seduta. Ora, ciascun senatore - come lei ben sa - può presentare sulle dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio una sua proposta di risoluzione. Il Governo, Il Governo, da parte sua, ha diritto di porre la questione fiducia su qualsiasi strumento il Governo medesimo prescelga. È del tutto evidente che è data facoltà ai singoli senatori di presentare adesso una risoluzione, si presume, sulle dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio.

ma non può porre un limite alla presentazione di altre risoluzioni, da parte di altri colleghi, e non può porre un limite al Governo nello scegliere la risoluzione sulla quale porre la questione di fiducia.

se non al momento di un voto: su un articolo, su un emendamento o su una risoluzione. PRESIDENTE. Ma il voto ci sarà alla fine della discussione generale

nuova finestra"). Senatore Calderoli, lei ha tutto il diritto di chiedere e di auspicare che possa essere votata la sua risoluzione; ha tutto il diritto, ma il Governo, per prassi costante, non solo per interpretazione regolamentare, ha assoluto diritto di chiedere e di verificare la fiducia sulla base della risoluzione da esso prescelta

io manifesto naturalmente il consenso e la fiducia sull'oggetto che è al centro del nostro dibattito, cioè la relazione qui svolta dal Presidente del Consiglio. Il documento formale, sul quale la fiducia verrà posta, è altra cosa ed è soltanto il contenitore delle dichiarazioni svolte dal Capo del Governo onorevoli colleghi, signor Presidente, un obiettivo comune alla maggioranza e al Governo, rappresentato con chiarezza nella relazione del Presidente del Consiglio. Riprendo le sue parole. L'obiettivo comune è rappresentato dalle riforme, sulle quali abbiamo impegnato la nostra opera al momento della presentazione del programma dell'Unione, e dal rinnovamento del Paese che è il filo che guida il nostro impegno politico al servizio dell'Italia. Le soluzioni prospettate dal Presidente del Consiglio sono, nell'ambito del programma, oggi, di fronte agli avvenimenti più recenti e al livello raggiunto dal dibattito politico nel nostro Paese, «soluzioni concrete, realistiche, possibili» - ripeto ancore le sue parole - alle quali la maggioranza può

noi abbiamo un primo problema e un primo dovere politico verso il nostro elettorato e verso il Paese. Per dirlo nel modo più semplice, questo dovere politico è di preservare e salvaguardare il bipolarismo e le condizioni istituzionali dell'alternanza, che ha rappresentato nella storia della democrazia italiana un passo avanti e una conquista. Il Il bipolarismo è strettamente legato ad un principio fondamentale proprio del nostro modo di intendere la politica, cioè il principio di responsabilità. Il cittadino vota su un programma, su uno schieramento, su un'ipotesi di Governo. Chi governa, chi è eletto risponde di fronte al cittadino che ha votato. Non c'è una delega in bianco, non c'è la continuità di un potere inamovibile. Invece, l'articolarsi di rappresentanze che esprimono le articolazioni della società, nelle quali si manifestano punti di vista plurali.

Questo è il bipolarismo, questa è l'assunzione di responsabilità che deve guidare il nostro impegno politico. L'impegno per il bene comune richiede, signor Presidente, questa assunzione di responsabilità.

Sì, esso c'è ed è giusto che ci sia. Ciascuno ha la propria storia, e non vuole rinunciare ad essa. Ciascuno ha la propria fisionomia culturale e politica, e per questo ci confrontiamo. Il bene comune richiede, però, non soltanto lo spirito di parte - che c'è e deve esserci perché è scritto nella storia - ma anche la disponibilità al confronto e alla ricerca dell'intesa. questa disponibilità nella relazione del Presidente del Consiglio. È una disponibilità che la maggioranza condivide ed in particolare essa è stata più volte riaffermata dal Gruppo dell'Ulivo. Noi dobbiamo - io credo - individuare i temi sui quali è necessario un intervento riformatore, sui quali è possibile perseguire obiettivi di riforma, attraverso un confronto ed anche un'intesa con quella parte dell'opposizione che ci appare più ragionevole e più disponibile al dialogo. La sintesi, che ci è stata proposta dal presidente Prodi e che non copre tutto l'ambito delle materie cui si riferisce il programma, indica anche alcuni terreni sui quali si può ricercare il confronto e l'intesa. Questo, infatti, è parte di un bipolarismo civile, nel quale non vi è soltanto lo spirito di fazione, ma vi è anche la ricerca di obiettivi comuni per le diverse parti che compongono il sistema politico. la politica internazionale, il presidente Prodi ha riproposto qui le linee di politica estera che erano già state limpidamente esposte mercoledì scorso dal ministro D'Alema: il primato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, la vocazione dell'Italia a dare forza al diritto internazionale, la scelta europea, il significato della missione in Libano e del ruolo di promotrice che ha avuto l'Italia per quell'intervento pacificatore. Il presidente Prodi ha sottolineato un rischio e ha posto un problema con il quale dovremo fare i conti nei prossimi mesi. Le scelte della *leadership* iraniana hanno creato una grave tensione, ma, proprio per questo, noi dobbiamo fare tutto il possibile perché le soluzioni siano negoziali, per evitare che si ricorra ad una soluzione militare, all'uso della forza. Ancora il dogma della guerra preventiva rischia di dominare l'orizzonte della politica internazionale, con risultati che, come dimostra l'esperienza, non possono essere positivi. E ancora: la solidarietà e la cooperazione internazionale. Anche questo è un tema sul quale è possibile trovare un'intesa; è possibile, cioè, che l'Italia esprima una politica largamente condivisa da questo Parlamento. Il presidente Prodi ha, poi, toccato alcune questioni di politica interna e di politica istituzionale che hanno particolare rilievo, a partire dalle liberalizzazioni. C'è un significato riformatore nel progetto di liberalizzazione di cui il Governo è portatore. dimostra la volontà di rompere le cristallizzazioni sociali che bloccano o impediscono la crescita, lo sviluppo, la conquista di una piena dignità delle persone. Questo è il significato di una politica di liberalizzazione, correttamente intesa come promozione delle possibilità e delle occasioni di vita degli individui, come rottura dei privilegi e delle cristallizzazioni sociali. Vi sono, poi, altri aspetti che sono importanti per il programma del centro-sinistra e che voglio qui richiamare: la politica del lavoro e la politica della casa, del diritto all'abitazione. Tante volte ascolto stucchevoli tiritere sulla politica a sostegno e in difesa delle famiglie. Ma cosa c'è di più importante per il sostegno alle famiglie che garantire il futuro ai giovani, il lavoro e la casa ai giovani? Dobbiamo realizzare assieme queste cose, presidente Prodi. Lei, credo, sappia qual è l'impegno e la dedizione del nostro Gruppo parlamentare alla coesione dell'Unione. Noi ci impegniamo nel lavoro parlamentare a far sì che le proposte del Governo possano trovare consensi anche al di là della maggioranza che ha vinto sul filo di lana le elezioni nella primavera del 2006.

di captare qualche ulteriore voto. La vera storia della sua crisi, però, parte da quelle 280 pagine che lei ha scritto circa un anno fa;

il centro-destra, mandiamo a casa Berlusconi. Bene, riuscito l'intento, adesso ne paga lo scotto, Presidente: ognuno ha preteso di realizzare ciò che aveva voluto leggere in quei 280 fogli così poco chiari del suo programma e, così, scoppiano casi a ripetizione, a cascata: la TAV, Vicenza, l'Afghanistan e, per ultimo,

le politiche della sicurezza e della difesa, che rappresentano l'immagine del nostro Paese all'esterno, e le politiche della famiglia. Su queste tematiche non è consentito andare a raggiera, come questo Governo ha dimostrato.

quello che a noi fa un po' specie, quello che ci risulta molto strano è che il Governo non è caduto su un tema politico, ma è caduto sulla superbia

essere corretto ed onesto intellettualmente e ammettere che vi è continuità nei rapporti con l'Alleanza Atlantica sul fronte delle missioni estere. No, questo non si può, anzi non si deve assolutamente dire; infatti, il *leit motiv* del vostro del vostro governare è stata la discontinuità: avete coniato un nuovo termine per fare le stesse cose che si facevano prima, ma chiamandole, etichettandole in un'altra maniera. In questo modo, le missioni militari sono diventate missioni di pace;

probabilmente occuperanno una mezza paginetta. Il passo che lei ha compiuto probabilmente è stato grande, ma non vi è stata maggiore chiarezza nel determinare l'azione di Governo.

Leggiamo anche di un ministro, Mastella, che si affianca a Dini ed esultano perché sono stati accantonati i Dico dal nuovo programma di Governo. Lo stesso giorno, sullo stesso giornale, due ministre,

parlamentari. In sostanza, le riserve mentali sul suo programma continuano ad esserci come prima, anzi adesso ve ne sono addirittura forse più di prima. Questa ambiguità voluta, presidente Prodi, noi non ve la possiamo perdonare. La sua maggioranza non ha solo problemi che potremmo definire di difetto di numeri; il vero difetto è di coesione: questo manca al suo Governo. Presidente, che figuraccia poi quel punto 12, che recita, più o meno, che l'ultima parola spetta al *premier*. Pare così naturale

Probabilmente significa che nell'Unione, finora, non è stato così. Presidente, lei si è dichiarato prigioniero della struttura che lei stesso ha costruito.

ha sempre affermato che la sua investitura derivava dalle primarie e questo dovrebbe essere fonte di legittimità sia politica che di ruolo, senza doverlo affermare in un punto programmatico.

Presidente, non ci sono soluzioni tecniche che risolvono problemi politici. Il nostro consiglio è di non accanirsi a prendere in giro tutto il Parlamento; concluda in fretta questo teatrino, o pantomima che dir si voglia e, secondo noi, potrà mantenere dalla sua almeno una parte delle persone ancora ragionevoli del nostro Paese.

il 18 maggio 2006 in quest'Aula ho dichiarato la mia fiducia a lei e al suo Governo, fiducia legata alla stima per la sua persona, alla condivisione delle linee generali del programma di legislatura, all'attenzione da lei garantita nei confronti delle autonomie speciali e della mia Regione, la Valle d'Aosta. Da quel giorno il mio sostegno è stato leale, serio e responsabile, sempre. Come Gruppo per le autonomie abbiamo apportato ai lavori un contributo costruttivo, improntato al dialogo con tutti, anche con i colleghi dell'opposizione. Ci siamo trovati di fronte ad una grande responsabilità, avendo ogni singolo nostro voto un peso politico determinante, ma le difficoltà che sono emerse in questa Aula non sono certo da ascriversi alle posizioni dei membri del nostro Gruppo. Per parte mia, unico rappresentante della Regione autonoma Valle d'Aosta, Vallée d'Aoste, in Senato, ho assistito con preoccupazione allo spettacolo della politica in questi primi mesi di legislatura, ma anche con il disagio di chi, per anni, è stato confrontato all'imperativo di assumere decisioni concrete delle quali dover rispondere alla propria comunità. componenti dell'Esecutivo che si sono dissociati dalle posizioni del Governo, nei dibattiti televisivi, con articoli di stampa, nelle manifestazioni di piazza non sempre hanno testimoniato della coesione necessaria per affrontare un percorso politico sereno. Abbiamo apprezzato, signor Presidente, la sua relazione in particolare sulla politica estera, sulle iniziative a favore della famiglia ed abbiamo, signor Presidente, apprezzato in modo particolare il riferimento specifico alle autonomie speciali e alle minoranze linguistiche. Oggi siamo chiamati ad esprimere nuovamente la nostra fiducia, per lo stesso senso di responsabilità e spirito di coerenza siamo disponibili a farlo: responsabilità e coerenza che chiediamo però anche al Governo tutto ed alla maggioranza che lo sostiene. Al Presidente della Repubblica, che ringraziamo ancora per l'attenzione dimostrata verso le autonomie storiche e le minoranze linguistiche, abbiamo riconfermato la nostra disponibilità in tal senso. Abbiamo, però, anche espresso al Capo dello Stato le nostre preoccupazioni, per la sensibilità distratta rivolta alle autonomie speciali percepita in questa prima fase di legislatura. Non possiamo accettare il continuo manifestarsi di tentativi volti a cancellarle o ad affievolirle. Le specialità devono essere salvaguardate, promosse e valorizzate. II generale rafforzamento delle Regioni a Statuto ordinario ci vede d'accordo, così come concordiamo con le iniziative che mirano a dare innovato slancio alle autonomie locali. ciò dovrà avvenire sempre nel pieno rispetto delle prerogative costituzionali, statutarie e ordinamentali delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome. Chiediamo il rispetto assoluto delle nostre specificità e della nostra autonomia politica e finanziaria; chiediamo che i rapporti con lo Stato siano improntati a pari dignità, leale collaborazione, condivisione degli obiettivi e partecipazione nelle scelte; chiediamo l'intangibilità degli statuti speciali e della loro forza, per le cui modifiche sarà essenziale addivenire alla codifica di una procedura di intesa; chiediamo che le Commissioni paritetiche - vitali per le nostre autonomie - siano pienamente operanti e che il Governo si esprima senza ritardo sulle disposizioni attuative. Chiedo, dunque, al Governo una precisa attenzione su questo punto. E' poi necessario valorizzare il ruolo e le attività delle Regioni e delle Province autonome a livello europeo affinché l'Europa non diventi lo strumento occulto per svilire le articolazioni substatali della Repubblica. Occorre anche incentivare le forme di collaborazione e di cooperazione interregionale (penso alle Regioni frontaliere e alle Regioni di montagna che necessitano di trovare una loro specifica collocazione e una particolare attenzione in Italia e in Europa).

Per quanto attiene al programma concordato in relazione alla Valle d'Aosta, abbiamo consegnato un documento che contempla le problematiche di rilievo e sulle quali chiedo l'attenzione del Governo. Non vogliamo privilegi, ma solo il riconoscimento e la tutela dei nostri diritti, la conferma che situazioni diverse vengano considerate con approcci diversi, rifuggendo ogni logica di omologazione,

Presidente, onorevoli senatrici e senatori, onorevole Presidente del Consiglio, ho apprezzato l'intervento con cui ha rinnovato l'ipotesi

ricordate, proprio perché abbiamo assistito a forme inedite di aggregazione, di lotta di cittadinanza e di territorio. E ho apprezzato ancora di più i richiami alla necessità di una lotta alla precarietà della condizione di lavoro. il Ministro del lavoro ricordava che in questi mesi sono stati trovati 50.000 lavoratori in nero nell'edilizia, che segnano la drammatica condizione e la storia del lavoro concreto nel nostro Paese, la storia, appunto, del lavoro vivo. Il lavoro continua ad essere, oggi, il collegamento fondamentale tra destini individuali e collettivi. Esso continua ad essere un requisito essenziale, non rinunciabile, per la partecipazione alla società. Nessuna protezione sociale può compensare la menomazione di diritti di cittadinanza dovuta all'assenza del lavoro o prodotta dalla precarietà, definendo così processi di vera e propria esclusione. Per questo ho anche apprezzato il richiamo all'aumento delle pensioni minime, seppure è nota la posizione di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, in perfetta sintonia anche con le grandi organizzazioni sindacali del nostro Paese,

al nostro Paese altri sistemi pensionistici e sociali - che il nostro è un sistema di Stato sociale ancora basato sul lavoro e sui contributi dei lavoratori, mentre in gran parte

prosecuzione dell'azione di Governo di questo Paese, una possibilità perché le classi sociali economicamente subalterne trovino una speranza, una possibilità di cambiare profondamente la loro condizione di vita. Diceva un grande dirigente del movimento operaio, una grande figura del sistema politico del Novecento, lontano lontano dalla mia cultura politica, Pietro Nenni: la storia della sinistra è storia delle occasioni perdute. Noi non vogliamo perderne altre, vogliamo invece che questo Governo, che ha innovato anche sul piano della costruzione del programma, sul terreno della ricerca di nuovi spazi di democrazia e di rappresentanza, come prima cercavo di ricordare, vada avanti e costruisca per quelle classi sociali a cui facevo riferimento (i giovani, chi è in condizioni di precarietà, chi vive del proprio lavoro, tante famiglie che faticano a raggiungere la fine del mese), nuove del mese), nuove prospettive e nuove possibilità. Per questo, convintamente, sosteniamo che c'è la necessità di proseguire questa esperienza di Governo, che ci sembra significativa.

poteva e doveva essere affrontata attraverso l'iniziativa su tre terreni. Il primo terreno è quello dei contenuti dell'azione di Governo su cui la crisi era precipitata, con particolare riferimento - ma come lei, presidente Prodi, ha giustamente detto questa sera, non soltanto con riferimento a questo - alla politica estera con la bocciatura della mozione di maggioranza. Il secondo terreno è quello del rafforzamento e del consolidamento della *leadership* della compagine di Governo e della coalizione dopo una troppo lunga fase di aperta competizione, quando non di scontro, tra le diverse componenti del centro-sinistra. Il terzo è quello della ristrutturazione del centro-sinistra stesso e dei suoi partiti laddove la presenza dei Gruppi dell'Ulivo, pure importantissima e per alcuni delicati passaggi decisiva ai fini della tenuta del Governo e della coalizione, non appare sufficiente a garantire all'intera coalizione uno stabile equilibrio, specie nel rapporto tra centro-sinistra riformista e sinistra antagonista. Con il suo discorso, signor presidente Prodi, lei ha affrontato con determinazione e, a mio avviso, con esiti positivi, due dei tre campi d'iniziativa cui si trovava confrontato. Il terzo, quello dell'innovazione dei soggetti politici del centro-sinistra e la conseguente ristrutturazione dei loro rapporti, non poteva e non doveva essere oggetto della sua iniziativa in quanto Presidente del Consiglio. È in atto nella vasta area del riformismo di centro-sinistra una discussione sul progetto che va sotto il nome di Partito democratico. Non intendo occuparmene in questo intervento, se non per sottolineare che, a mio avviso, anche la crisi di Governo segnala l'urgenza di una forte accelerazione: senza un grande partito riformista a vocazione maggioritaria, che raccolga la gran parte dei consensi necessari al centro-sinistra per prevalere sul centro-destra, l'intera coalizione non possiede tutta la forza politica necessaria a guidare l'Italia nell'immane sforzo di cambiamento che solo può evitarne il declino. Sui due terreni che le erano propri in quanto Presidente del Consiglio, lei si è mosso con efficacia in questi giorni, e anche nel suo discorso di questa sera, nella direzione dell'auspicato rafforzamento. Delle posizioni in tema di politica economica e sociale che lei ha richiamato voglio sottolineare, in primo luogo, la piena coerenza con le linee del Documento di programmazione economico-finanziaria, presentato dal Governo a giugno. Obiettivo unificante: la crescita significativa e duratura nel tempo. Per conseguire questo obiettivo sono tre le mosse fondamentali di politica economica: la prima, già portata a termine, è la riduzione del cuneo fiscale e contributivo sul lavoro; la seconda, le liberalizzazioni e la riduzione del volume globale del debito. Per le prime parlano i disegni di legge su cui lei rinnova questa sera l'impegno del Governo e chiama la maggioranza a superare ogni incertezza: entro luglio, quei disegni di legge dovranno diventare legge e dovranno essere emanati gli atti amministrativi previsti (penso alla separazione proprietaria di SNAM Rete gas dall'ENI) dalla legislazione vigente. Per la riduzione del volume globale del debito, il punto 7) del dodecalogo supera i limiti della stessa legge finanziaria, laddove rinnova l'impegno a ridurre la spesa pubblica sia in generale (e l'impegno a unificare gli enti previdenziali è in questo quadro, secondo me, assai significativo) sia con specifico riferimento ai costi della politica. Infine, la terza mossa: investimenti in infrastrutture materiali e immateriali. La legge finanziaria definiva già una svolta laddove, dopo sei anni consecutivi in cui ciò non era accaduto, autorizzava una spesa in conto capitale più elevata del livello del *deficit*. Il bilancio 2007, colleghi, rispetterà quella che gli economisti chiamano la regola aurea, ma da sei anni ciò non accadeva nel bilancio pubblico italiano. Ma oggi lei qualifica e specifica l'orientamento suo e del Governo: dopo i porti, priorità cui cui si è mirato per le infrastrutture nella legge finanziaria, ora i grandi corridoi europei e i rigassificatori. È stato detto e scritto che si tratterebbe di impegni generici: mi sembra vero esattamente il contrario. Sono obiettivi difficili, come sappiamo, anche per questa maggioranza, ma sono obiettivi molto precisi. A proposito di politiche del lavoro e con particolare riferimento alle politiche volte a ridurre la precarietà dei rapporti di lavoro, ho letto di giudizi di insoddisfazione, il tema sarebbe assente. In tutta franchezza, non riesco a concordare con questo giudizio. Il Governo e la maggioranza hanno appena finito di licenziare una legge finanziaria che contiene, nell'ordine, le seguenti misure. Primo: la riduzione di ben tre punti di cuneo fiscale e contributivo sul lavoro beneficia esclusivamente le imprese che hanno rapporti di lavoro a tempo indeterminato: esclusivamente, colleghi, non prevalentemente o prioritariamente. Secondo: Secondo: il ricorso a contratti atipici viene scoraggiato con forti aumenti delle aliquote contributive per questo tipo di lavoratori. Non c'è, infatti, alcuna ragione economica per la quale questo lavoro debba costare meno di quello stabile. Terzo: per le lavoratrici atipiche si avvia l'istituto dell'indennità di malattia e di maternità, mentre l'assunzione di una lavoratrice nel Sud darà luogo ad un forte vantaggio per l'impresa rispetto all'assunzione di un lavoratore maschio. Quarto: gli enti locali, dove si concentra ciò che rimane delle cosiddette collaborazioni coordinate e continuative, sono autorizzati e aiutati finanziariamente a stabilizzare i rapporti con questi lavoratori. Non basta? Certo, ma quel che c'è è davvero molto e quel che non c'è ancora, un sistema universale di ammortizzatori sociali capace di coprire tutti i lavoratori italiani in difficoltà, potrà essere realizzato se saremo capaci di un effettivo riequilibrio nella spesa pubblica a favore di chi ha di meno, di chi sa di meno e di chi può di meno, ma non per ribadirlo nella sua condizione di debolezza, assistendolo un po' meglio, ma per aiutarlo davvero a farcela da solo nel mercato. Infine, lei chiede ai Partiti dell'Unione di riconoscerle, signor Presidente del Consiglio, l'ultima parola, quella decisiva in caso di contrasto. Una pretesa, la sua, perfettamente coerente con il carattere che la forma di Governo è venuta assumendo anche nel nostro Paese, secondo il modello delle democrazie competitive di tipo europeo. Dunque, una pretesa cui i Partiti dell'Unione debbono - come hanno fatto - rispondere convintamente sì. A questo proposito, il limite è dato dal contrasto fortissimo tra quella centralità della *premiership*, cui ho già fatto riferimento e di cui la sua richiesta è espressione, e la logica di fondo della legge elettorale: dove la prima reclama disciplina e coesione, la seconda spinge alla frammentazione e alla competizione interna allo schieramento. È una contraddizione che andrà affrontata nell'interesse non di questo Governo, ma del governo del Paese; ma va affrontata sulla base di una scelta precisa tra due opzioni possibili: il rafforzamento del bipolarismo attraverso l'innovazione nella struttura delle due coalizioni dei soggetti politici che le compongono e attraverso la scelta degli elettori tra due credibili offerte di Governo tra loro alternative; oppure la presa d'atto che l'Italia non è fatta per il bipolarismo, ma può essere governata solo da un partito di centro, ago della bilancia degli equilibri di Governo.

Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, la fiducia a un Governo non è un atto di fede, ma un atto politico. Del resto, il Governo non è il fine nelle forze politiche, ma uno strumento con cui le forze politiche si rapportano con la società e pensano e partecipano al governo di essa, al raggiungimento degli obiettivi che questa si pone. Ed è in questo quadro, con questo spirito, che mi sento e ci sentiamo sereni e convinti nell'apprezzare il discorso che lei, presidente Prodi, ha fatto; quello che ci ha proposto come occasione di verifica della fiducia del Governo e della coalizione. Mi pare che sia stato un atto di grande responsabilità e sensibilità politica quello da lei compiuto e un atto di saggezza quello del presidente Napolitano, che ha risposto positivamente alla dichiarata riconferma dell'impegno di tutte le forze dell'Unione. Voglio dire che questo impegno non riguarda soltanto le fasi ultime della gestione del Governo, ma un sedimentato politico che parte dalle primarie, dalla costruzione del programma dell'Unione e dalla vittoria elettorale di stretta misura, ma comunque vittoria. Capisco che tutto questo possa determinare irritazione nell'opposizione, nell'opposizione, ma è meno comprensibile una serie di commenti e di comportamenti di alcuni vestali e sacerdoti del bipolarismo che in questi giorni si sono esercitati alla ricerca di intese trasversali di grosse coalizioni, di assemblaggi di volenterosi e radicali centristi.

gli elementi su cui si era determinato il confronto e lo scontro, sono spariti sostanzialmente. I giornali hanno parlato d'altro, i temi venuti all'emergenza sono altri; i senatori Turigliatto e Rossi, che con la loro - mi permetto di dire - improvvida arroganza di presentarsi come gli unici pacifisti rimasti nella sinistra, in qualche modo hanno tolto la scena agli altri pacifisti (che, per fortuna, in questa sinistra e in questo Paese ci sono e sono in tanti), hanno finito per essere sostanzialmente soggetti dei *talk show*. Ma c'è un punto su cui dobbiamo riflettere, che è stato determinato dalla distorsione politicista del dibattito di questi giorni, che ha fatto emergere una sorta di autonomizzazione della politica, che si è esercitata fuori e a prescindere dalla società, dalle sue contraddizioni, dai suoi bisogni. Il rapporto tra politica e società, che lei ha richiamato opportunamente e in più occasioni, e il rapporto tra società e istituzioni mi pare che siano il terreno su cui c'è lavoro per tutte le forze dell'Unione, per tutte quelle forze che costituiscono la ricchezza dell'Unione. E bene ha fatto non soltanto lei, ma anche il Presidente della Camera a riproporre questo tema in una recente intervista, perché in questa autonomizzazione della politica c'è il cinismo del potere,

cioè la costruzione di progetti politici a prescindere dalla concretezza dei rapporti sociali, dei consensi sociali, della faticosa costruzione delle condizioni che possono assentire ad una scelta di Governo, a faticose scelte di Governo. Penso che questa riflessione ci debba spingere tutti ad approfondire quel filo di ragionamento che lei ha proposto e che riguarda la stessa crisi della democrazia, perché quando parliamo della legge elettorale e della connessione che lei ha richiamato tra la legge elettorale e le misure d'intervento anche sulla seconda parte della Costituzione, credo che di questo, della struttura della democrazia, stiamo parlando. E allora, se è questo, mi chiedo: è è meglio o no, è indifferente per la politica se ci sarà più lavoro o meno lavoro, migliori o peggiori pensioni, se ci saranno - per dirla con Sandro Pertini - più trattori e meno carri armati? armati? Vorrei invitare tutti coloro che si sono esercitati in questi giorni (e anche oggi) nell'interpretazione dei 12 punti e ci hanno costruito editoriali e tavole rotonde a riflettere su un fatto, cioè che quando uno qualunque di questi 12 punti arriverà ad essere atto di Governo, si confronterà con la realtà, con i corpi intermedi della società plurale e articolata, si confronterà con quella gente normale, ma anche - mi permetto di dire - con chi, come noi di Rifondazione comunista, è disposto e interessato a interloquire e a discutere, ma non si lascia intimidire o condizionare dai toni ultimativi che usa qualcuno come la ministra Lanzillotta.

lei ha detto: «Non giudicatemi per quello che non avrò detto», ma francamente lei ha detto qui talmente poco che siamo costretti, in qualche misura, a doverci riferire a cose e a fatti detti in queste ore. ore. In queste ultime ore, gli esponenti del Governo e della sua maggioranza si affannano a comunicare all'opinione pubblica che il suo Governo otterrà sia la maggioranza numerica in quest'Aula (e questo era fuori discussione, visto l'apporto certo di quasi tutti i senatori a vita), sia la maggioranza dei senatori eletti, e per questo, signor Presidente del Consiglio, si dice che il suo Governo avrebbe una maggioranza politica. Mi permetto di obiettare che, se anche giungerà al suo Governo il voto del senatore Pallaro, come lui stesso ha annunciato in diverse interviste, siamo ben lontani da quella che si definisce una maggioranza politica. Il senatore Pallaro, infatti, dopo molti contrasti e molte riflessioni, ha deciso che voterà la fiducia al Governo, ma nulla ha lasciato intendere su come voterà successivamente sui singoli atti di Governo. Altri esponenti, poi, che fanno parte o dovrebbero far parte, presidente Prodi, della sua maggioranza politica, in quanto eletti sotto le bandiere della sua coalizione, hanno già detto che voteranno la fiducia, ma su atti fondamentali della politica del Governo voteranno contro: mi riferisco ai senatori Turigliatto e Rossi

Lei sta cercando di legittimarsi sulla base di uno strano sillogismo, secondo il quale non esisterebbe alternativa al suo Governo se non le elezioni, ma siccome alle elezioni non si potrebbe andare, perché la legge elettorale del Senato non funziona, non c'è alternativa al suo Governo fino a quando non si cambierà la legge elettorale. realtà, signor Presidente del Consiglio, è falso per un ragione molto semplice: perché se lei avesse ottenuto la maggioranza dei voti degli elettori la legge elettorale del Senato avrebbe funzionato e lei avrebbe potuto avere una maggioranza di senatori sufficiente a farle attraversare ogni temperie politica. Infatti, con qualunque altra situazione di voto,

La realtà è che non si può accusare la legge elettorale se lei e la sua alleanza non avete vinto le elezioni e, per quanto non vogliate piegarvi ai fatti e tentiate di piegare i fatti a vostro vantaggio, i fatti parlano in modo inequivocabile; dopo di che, signor Presidente del Consiglio, non regge la soluzione che lei avrebbe escogitato per risolvere i problemi della sua maggioranza e dei mancati voti che già si annunciano sui suoi provvedimenti: il suo dodecalogo poggia sulla sabbia,

tra le forze della sua maggioranza a provocare la caduta del suo Governo in quest'Aula, ma semplicemente il mancato voto di due senatori della sua maggioranza e un diverso orientamento di alcuni senatori a vita

quale lei dovrebbe finalmente prendere atto è che, non avendo vinto le elezioni, non può pensare di governare il Paese come se le avesse vinte e cercare di guadagnare tempo, rinviando alla riforma della legge elettorale la fine di un'esperienza fallimentare sul piano della coalizione politica.

Signor Presidente, svolgerò qualche notazione di tipo politico, perché incredulità e sgomento sono state le prime reazioni alle modalità con le quali questa crisi si è manifestata. Presidente Prodi, lei ha ricordato giustamente che siamo in un momento di crescita economica complessiva, a seguito anche di una finanziaria difficile e, per alcuni versi, coraggiosa. versi, coraggiosa. Ha ricordato inoltre che siamo in una fase di positivo protagonismo dell'Italia sullo scenario internazionale, dove stiamo dando un apporto decisivo alla politica di pace, anche in Medio Oriente. Eppure, proprio ora che il Paese sta cercando la misura per ripartire dentro la ricerca di un nuovo equilibrio sociale, si è consumata una crisi, a mio avviso in nome più del narcisismo delle idee che non di una politica che mira al bene del Paese. Ma forse non tutto il male viene per nuocere. Si sta infatti facendo chiarezza e si sta avviando un percorso politico che fa ben sperare che questo episodio appartenga al passato (seppur molto prossimo) e si possa considerare chiuso. Bene quindi ha fatto il presidente Prodi a stilare - come se questo fosse un richiamo prima di tutto alla responsabilità la famosa lista, che soprattutto nei primi nove punti contiene gli elementi fondanti e irrinunciabili, tratti dal programma votato dagli italiani, a cui dobbiamo lavorare con rinnovato vigore. Ma questo lavoro dovrà essere anche improntato, da parte del Governo, ad un rapporto proficuo con il Parlamento. È doveroso che l'Esecutivo avanzi le proposte di legge, ma è altresì corretto lasciare, nei termini della responsabilità dei paletti sopra citati, che il Parlamento possa esprimersi e, se necessario, introdurre adeguati correttivi. Quindi, per evitare possibili incidenti di percorso, la maggiore attenzione da parte del Governo al Parlamento potrebbe essere una condizione da aggiungere alla lista. E poi, con quale maggioranza con quale maggioranza politica fare questo lavoro? Questo appare ovvio: *in primis* con quella uscita dalle urne, ma più in generale, signor Presidente del Consiglio, con quella che voterà la fiducia. Quando abbiamo costituito l'Unione, come alleanza strategica e non raccogliticcia, sapevamo di dover usare grande capacità di mediazione ed una grande dose di responsabilità per arrivare ad un esito il più possibile condiviso nell'operato del Governo e nelle discussioni parlamentari. Capacità di mediazione e responsabilità devono quindi essere ancora i pilastri dell'agire politico e devono essere riscoperti e riutilizzati a piene mani contro ideologismi chiusi e personalismi, che sono i veri nemici della costruzione del bene comune. Solo così potrà reggere fino a fine mandato l'Unione e il Governo Prodi, cui essa è strettamente connessa: oggi non esiste Unione senza Prodi e non esiste Prodi senza Unione. Se è così, bisogna anche capire che la politica sta rapidamente evolvendo su un binario parallelo a quello della legge elettorale e che la capacità politica dell'Unione - e quindi del Governo - si dimostrerà anche nel saper cogliere questi mutamenti, nel non chiudersi a fortino dentro le proprie mura e nel saper aprire un dialogo senza paura con chi in Parlamento (soprattutto qui in Senato) dimostrerà di volerlo fare in termini di correttezza, senza snaturare la politica di questa alleanza (l'Unione) e senza snaturare l'attuazione del programma votato dagli italiani e rimarcato nella sua lista. Si dice che talora bisogna fare di necessità virtù. In questo caso, la necessità di stabilizzare la maggioranza politica qui in Senato sta permettendo un primo allargamento, segno di fiducia al Governo, ma anche di comprensione che, in un momento di delicata congiuntura internazionale, non possiamo lanciare il Paese verso l'ignoto di una paurosa crisi al buio. Caro presidente Prodi e cari colleghi, gli italiani, ma prima ancora la nostra responsabilità personale e politica, ci chiedono di andare avanti a governare, per accompagnare un Paese unito ed orgoglioso sulla via intrapresa dell'innovazione, della crescita economica, della credibilità internazionale e della sicurezza sociale. Quindi avanti, con sicurezza, per il bene del Paese!

una crisi politica su un aspetto fondamentale dell'attività di Governo. Non possiamo non chiederle ora se ritenga davvero risolta quella crisi se pensi che il voto di fiducia, ove espresso anche da una maggioranza che non computi i senatori a vita, possa garantire poi l'effettiva governabilità sui grandi nodi della politica internazionale, dell'etica pubblica, del nuovo modello sociale quale si realizza attraverso le politiche del lavoro, della famiglia, della previdenza, della competitività fondata su investimenti nella logistica e nell'energia. Tutti temi che lei ha prudentemente evitato, restando sui nodi reali che avrà di fronte a sé nell'attività di Governo assolutamente generico. In realtà, ciò che vogliamo sottolineare è che questa crisi investe la natura stessa della coalizione che intorno a lei si è organizzata. Questa coalizione, infatti - espressione, peraltro, di un processo che si era manifestato già nel corso di tutti gli anni Novanta - è stata realizzata sulla base di alcuni vizi fondamentali: la sottovalutazione di un fenomeno terroristico ideologizzato, che è figlio dell'estremismo antagonista, una certa dose di cinismo rispetto alle esigenze di riforma strutturale del Paese e, soprattutto, un bipolarismo esasperato che ha indotto la regola del «nessun confine a sinistra». Ora, credo che questa crisi abbia definitivamente evidenziato come in Italia vi sia una sinistra antagonista che non è abilitata a governare. Vi è una sinistra con caratteristiche rinvenibili anche in altri Paesi, ma che in altri Paesi non assume funzioni di Governo. Si tratta di una sinistra antioccidentale, esplicitamente tale, e come tale, non disponibile ad alcuna delle politiche che si muovono nel solco della nostra tradizionale politica estera. È una sinistra ostile all'economia di mercato e a tutte le sue espressioni, propugnatrice di un conflitto esasperato nelle relazioni industriali, perché convinta che il lavoro sia inesorabilmente l'epicentro di un virtuoso conflitto che avrebbe il pregio di muovere la storia. Una sinistra, infine, regressiva rispetto a tutte le esigenze di evoluzione del modello sociale, come le difficoltà che lei incontra sul tema della riforma previdenziale evidenziano. Come dicevo, anche in altri Paesi esistono espressioni analoghe, anche se non del tutto così ancorate ancora ad un'esplicita tradizione marxista, però queste non sono abilitate a governare. il caso del cancelliere Schröder che ha posto un esplicito confine a sinistra, perfino nei confronti di quella sinistra socialdemocratica rappresentata da Oskar Lafontaine, che non è certo - per quanto radicale - paragonabile alle caratteristiche di molta nostra sinistra interna. Ebbene, Schröder ha preferito non vincere le elezioni e poi accingersi ad una larga coalizione, piuttosto che comporre una coalizione incapace di governare e incapace di decidere sui grandi temi che sono comunque all'ordine del giorno di una grande democrazia industriale, impegnata, per un verso, nella transizione verso l'economia della conoscenza e, per un altro, sui grandi temi dell'equilibrio internazionale. Ecco, io credo che lei debba prendere atto della crisi irreversibile della sua maggioranza, della crisi cioè di aspetti fondanti della sua stessa coalizione. È importante che ne prenda atto perché lei ha soprattutto fondato l'equilibrio della coalizione, il modo quotidiano di governarla, rifacendosi proprio a quelle componenti più radicali che ho cercato - pur sommariamente - di descrivere come inadatte e inabilitate a governare. L'Italia ha bisogno di una nuova *conventio ad excludendum*, nuova, ma in realtà che si ricollega alla tradizione di ieri, perché riguarda ancora oggi, incredibilmente, i comunisti.

Come ormai è chiaro da riscontri e evidenze scientifiche, la crisi climatica sta subendo accelerazioni e va affrontata con misure incisive di riduzione dei gas di serra. Le conseguenze della crisi climatica sono già serie ma, in assenza di incisive misure di riduzione delle emissioni, diventerebbero drammatiche e irreversibili. L'Italia, come rilevato dalla Commissione europea, sarebbe fra i Paesi mediterranei più colpiti. Il nostro territorio ne verrebbe sconvolto e le conseguenze per l'economia e suoi settori chiave, come turismo e agricoltura, sarebbero pesantissime.

cogliendo anche l'opportunità, che l'Unione Europea definisce di una nuova rivoluzione industriale, richiesta e promossa dal futuro a basse emissioni di carbonio. In questa nuova rivoluzione industriale siamo pesantemente in ritardo. Mentre l'Unione Europea propone, a livello internazionale, un obiettivo di riduzione dei gas di serra entro il 2020 e dichiara che anche in mancanza di un accordo internazionale su tale obiettivo assumerà unilateralmente un impegno di riduzione del 20

che, se dovessimo pagare con acquisti di diritti di emissione, corrisponderebbe ad una spesa annua stimabile in almeno 1,5 miliardi di euro. Nei trasporti, le emissioni di gas di serra sono cresciute, dal 1990 al 2005, del 23 nella produzione di energia elettrica, del 21 per cento. La crescita maggiore di emissioni negli ultimi anni si è verificata proprio nel settore della produzione di energia elettrica con ben 10 milioni di tonnellate di CO2 di maggiori Per ragioni di tempo, mi limito ad alcune considerazioni sulle energie rinnovabili, che sono cruciali, come anche lei ha ribadito, per affrontare la crisi climatica. Le energie rinnovabili in Italia non crescono. Nel 2000 abbiamo prodotto 51,4 terawatt/ora con fonti rinnovabili, nel 2005 ne abbiamo prodotto 50 a causa della riduzione della produzione idroelettrica, non compensata dalla modestissima crescita delle nuove fonti rinnovabili. La percentuale della quota di fonti rinnovabili sul consumo interno lordo di energia elettrica è così calata dal 16 per cento nel 2000 Ricordo che la Germania nello stesso periodo ha, invece, raddoppiato la propria produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. L'Unione ha assunto nel proprio programma elettorale l'obiettivo della direttiva europea del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2010 con fonti rinnovabili. Supponiamo che le misure, buone e adottate per migliorare il risparmio e l'efficienza energetica, fermino la crescita dei consumi elettrici a 360 terawatt/ora, cioè il consumo attuale, al 2010. L'obiettivo del 25 per cento richiederebbe una produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di 90 terawatt/ora, cioè 40 in più di quelli prodotti nel 2005. Contando l'effetto del sistema di incentivazione vigente, si arriva ad una crescita modesta, meno di un terzo dell'impegno necessario per raggiungere il 25 Sottolineando con grande favore l'impegno da lei ribadito per le fonti rinnovabili, ritengo che dobbiamo produrre uno sforzo straordinario, già nei prossimi mesi, per realizzare una riforma del sistema delle fonti rinnovabili in Italia, riforma indispensabile per raggiungere l'obiettivo del 25 per cento ma anche per fare fronte agli impegni di Kyoto. Per questo impegno straordinario per lo sviluppo delle energie rinnovabili penso sarebbe molto utile e importante anche un impegno dell'opposizione. I nodi di questo impegno (tra l'altro proposti all'esame del Senato) a mio parere sono cinque. la riforma del sistema di incentivazione di tutte le fonti rinnovabili (idroelettrica, eolica, solare, biomasse, biogas, geotermia) perché con il sistema attuale si resta molto lontani dall'obiettivo del 25 occorrono norme che assicurino più efficace e rapida connessione e dispacciamento delle rinnovabili. Inoltre, troppe Regioni e Comuni pongono ostacoli allo sviluppo delle fonti rinnovabili. L'obiettivo del 25 per cento va assunto come vincolante, con un programma concordato tra lo Stato e le Regioni, con obiettivi conseguenti, ripartiti fra tutte le Regioni. Per chi non opera per tali obiettivi, andrebbero previsti poteri sostitutivi con la nomina di commissari *ad acta*. È necessaria, infine, una riforma delle procedure di localizzazione e di realizzazione degli impianti per le fonti rinnovabili: quelle vigenti sono troppo lunghe, incerte, spesso inconcludenti. E' indispensabile anche il potenziamento del supporto tecnico Il cambiamento del sistema energetico è tecnicamente ed economicamente fattibile, ma, come faceva notare Bill Clinton alla Conferenza di Montréal citando Macchiavelli,

finestra") *(FI)*. Signor Presidente, colleghi senatori, signor Presidente del Consiglio, abbiamo ascoltato le sue dichiarazioni, con cui ha illustrato le priorità

un impegno preciso per il proseguimento della missione in Afghanistan e un impegno preciso per la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione. Su questi due argomenti qualcuno, evidentemente, alla fine dei giochi resterà ingannato.

di Governo. Francamente, non credo che questo succederà, anche perché sappiamo che la maggioranza in generale del Parlamento è certamente favorevole a tale missione. Probabilmente, allora, resteranno ingannati gli elettori che hanno votato per certi partiti, che sulle missioni militari all'estero - e in particolare sulla missione in Afghanistan - si sono pronunciati contro in modo estremamente forte e costante. Abbiamo sentito in quest'Aula soltanto la settimana scorsa, quando vi è stato il dibattito sulle dichiarazioni del ministro D'Alema, affermazioni, anche sconcertanti, ma certamente coerenti con quanto viene detto nelle manifestazioni e con quanto è stato detto nella campagna elettorale. Abbiamo sentito enunciare le gloriose vittorie

Nei suoi impegni, signor Presidente del Consiglio, c'è invece il proseguimento della missione in Afghanistan. Non è menzionato, ma è evidente che, non essendoci nulla di nuovo, si proseguirà con l'ampliamento della base militare di Vicenza.

fortemente, in modo così convinto, con argomenti anche molto forti, si sono pronunciati contro questa missione, che abbiamo sentito definire come missione di guerra, come missione di aggressione. Abbiamo sentito definire le basi

Pure *leader* di partito, come l'attuale ministro Pecoraro Scanio, sono andati in Val di Susa a dare il loro pieno e incondizionato appoggio a chi, sia della Val di Susa che proveniente da fuori, manifestava contro quella linea ferroviaria. Va anche ricordato che la maggior parte di loro si oppongono in ogni caso. Si dice che si realizzerà questa linea ferroviaria,

dunque vorrà dire aver ingannato tutti coloro che hanno votato certi partiti perché si sono schierati esplicitamente contro questa opera infrastrutturale, quasi come una bandiera;

oggi il nostro Paese non ha bisogno di un Governo stabile purchessia, ma ha bisogno di questo Governo, del Governo Prodi. Ne ha bisogno perché è questa la soluzione più avanzata per il rilancio dell'economia, per l'ampliamento dei diritti, per la costruzione di un mondo di pace. Credo sia necessario riportare il dibattito febbrile di questi giorni alle sue giuste proporzioni. C'è una domanda di concretezza che viene dal Paese al quale dobbiamo saper dare una risposta non evasiva né sfuggente. La crescita dell'economia oggi in atto è un fatto importante che ci consente di affrontare con serenità il vero nodo della nostra azione, quell'idea di sintesi felice tra diritti e benessere. Tenere insieme equità e sviluppo è stato fin dall'inizio il tratto distintivo del programma di Governo dell'Unione ed è questa la sfida da cui dobbiamo ripartire. Di fronte ad una lettura strumentale che alcuni fanno di noi, cioè del centro- sinistra, come fossimo un'alleanza costituita da moderati e radicali l'un contro l'altro armati, rispondiamo con il passaggio di oggi e di domani, dando il segno chiaro dell'unità della nostra coalizione, un'unità fondata su una seria analisi dei problemi e una precisa azione politica conseguente. Ci affideremo ancora a quel patrimonio grande che è il programma dell'Unione fatto non solo di 281 pagine, ma della passione e della competenza di centinaia di uomini e di donne che lì hanno messo le speranze che poi sono state premiate. Dimostreremo la nostra unità con il voto di fiducia domani e, giorno dopo giorno, continueremo a dimostrarla con la costruzione di un'economia più libera, la riforma dei luoghi del sapere, la lotta contro il precariato, la presenza autorevole del nostro Paese in Europa e nel mondo. Non possiamo nascondere il nostro rammarico, il mio rammarico, per quanto avvenuto in questa stessa Aula la settimana scorsa, un rammarico profondo che ha coinvolto non solo noi ma milioni di cittadini, rammarico e smarrimento da cui sono sorte poi forti dimostrazioni di sostegno. Anche da qui ricaviamo l'incoraggiamento a rinnovare la nostra fiducia al Governo Prodi. Prendiamo atto che il Presidente del Consiglio ha ritenuto, con un chiaro atto politico, di rassegnare le dimissioni nelle mani del Capo dello Stato, ma non possiamo nascondere di essere rimasti colpiti dal fatto che questo sia avvenuto sulla politica estera, proprio sul terreno dove oggi l'Italia ha acquisito un ruolo più forte, più autonomo e più autorevole. Citiamo solo tre dati che non possono essere sottaciuti: il rifiuto di ogni azione unilaterale, che ha portato innanzi tutto al ritiro dei nostri soldati dall'Iraq; il coraggio di guidare una forza di interposizione in Libano che sia realmente terza e a salvaguardia dell'incolumità dei civili; un approccio chiaro e risoluto perché l'annoso, drammatico conflitto tra israeliani e palestinesi si risolva con due Stati liberi e sovrani come da anni auspichiamo. Ecco da dove nasce l'autorevolezza cui facevo riferimento e che è certificata dal larghissimo consenso con cui oggi sediamo nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Nonostante tutto questo, proprio sulla politica estera sono sorte le difficoltà che oggi registriamo. Questo momento di crisi può avere due esiti opposti: o togliere slancio alla nostra azione, spingerci a galleggiare in attesa di non si sa che cosa, come si augurano molti esponenti dell'opposizione, oppure farci ripartire con più forza, più convinzione, più unità, ciascuno consapevole della propria responsabilità ma soprattutto dell'opportunità storica rappresentata da questo Governo, perché dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista, di questo si tratta, di un'opportunità storica che solo una vera e propria cecità politica potrebbe negare e noi ciechi non siamo, lo diciamo proprio a partire da quei 12 punti proposti dal presidente Prodi e sottoscritti dalla maggioranza. Come non cogliere che lì sono indicate le grandi questioni che determineranno la possibilità di futuro della nostra comunità nazionale? Come non cogliere, per esempio, la scelta di porre subito dopo la politica estera il sapere, la ricerca, l'innovazione come assolute priorità? E allora ripartiamo da qui, da una nuova consapevolezza sulla centralità del sapere nella nostra società. Quando abbiamo affrontato la sessione di bilancio, nei mesi passati, abbiamo spesso sentito parlare di una finanziaria senz'anima; oggi, con i 12 punti, si conferma la cifra della nostra maggioranza: il sapere e l'innovazione l'unica leva che consentirà tanto alle nostre imprese di essere competitive in uno scenario internazionale sempre più aggressivo, quanto ai nostri giovani di avere una speranza, di non andare incontro ad una vita precaria. Vorremmo che fosse chiaro allora, che non stiamo insieme solo perché non tornino le destre al Governo; l'anomalia della destra italiana ci è nota a partire dal pesantissimo conflitto d'interessi che la caratterizza e altrettanto chiare ci sono le conseguenze delle scelte del precedente Governo sulla vita degli italiani, l'impoverimento delle classi più deboli, partecipazione alla guerra permanente e preventiva, fino addirittura all'adesione e all'ideologia dello scontro di civiltà. Stiamo insieme anche perché solo a questa coalizione è concessa una sintesi nuova ed alta: coniugare diritti e crescita, opportunità e sviluppo, uguaglianza e libertà. Per noi questo vuol dire anche rafforzare i diritti, riformare il sistema del *welfare*. Alcuni capitoli: l'urgenza di aumentare il reddito degli incapienti e la necessità di garantire il diritto alla casa per tutte e per tutti; la costruzione di una rete vera di asili nido che consenta alle donne di accedere e mantenere il lavoro. Chi ha l'idea distorta di un conflitto tra moderati e radicali vedrà che questi sono obiettivi di tutti noi, di tutto il centro-sinistra. Oggi, di fronte a queste sfide, siamo chiamati a confermare la forza della nostra maggioranza, ma è utile sottolineare come la maggioranza politica non sia mai venuta meno. Non si tratta di sottacere quello che è successo o di usare l'alibi dell'incidente di percorso; si tratta, invece, di avere la piena consapevolezza del frutto avvelenato lasciatoci da chi oggi siede nei banchi dell'opposizione. Con questa legge elettorale non è garantita la governabilità del Paese e questo è un problema di tutto l'arco costituzionale, maggioranza e opposizione. Siamo convinti che, salvaguardando rappresentatività e bipolarismo, sia possibile trovare in Parlamento un'opzione forte e chiara capace di garantire questo principio di governabilità, ma lo diciamo con umiltà. L'ingegneria elettorale non può sostituire la politica, lo sforzo quotidiano di far prevalere l'interesse generale su quello particolare, la fatica della sintesi. Per noi il Governo guidato da Romano Prodi, il nostro Governo, è questo: il valore della politica. Già importanti risultati abbiamo costruito in questi mesi: un rinnovato impegno di pace in politica estera, una rigorosa azione contro l'evasione fiscale, misure di contrasto della precarietà; per la scuola è stato avviato un processo di rinnovamento e qualificazione, basti pensare all'innalzamento dell'obbligo a sedici anni. Di fronte a questi risultati non credo che la società italiana potrebbe accettare un periodo di stasi o soluzioni pasticciate. La politica ha il compito oggi di dare indicazioni, sostenere e accompagnare il processo di crescita in atto. l'Italia non può permettersi di diventare il fanalino di coda dell'Europa. La soluzione rappresentata dal presidente Prodi, invece, è l'unica possibile ed è la più avanzata ed equilibrata. Il rinnovo della fiducia al Governo dell'Unione accentua, dunque, le prerogative e la centralità del Parlamento, incoraggia a proseguire con determinazione l'azione politica per la giustizia e lo sviluppo,

Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, lei giustamente nel suo intervento ha posto in primissimo piano, con priorità assoluta, il discorso relativo alla politica estera e di difesa, argomento sul quale, tra l'altro, è stata smentita la politica del Ministro degli esteri e quella del Ministro della difesa proprio in quest'Aula, dando vita alla crisi nella quale vi state dibattendo. Debbo anche dire che, in realtà, avete smesso di parlare di discontinuità e questo è molto positivo. Finalmente - era ora - avete smesso di parlare di discontinuità

incorrendo anche in parecchie inesattezze. Vi ricordo che tutte le operazioni di pace alle quali l'Italia ha partecipato sono state operazioni multilaterali; non avete inventato proprio nulla.

sotto l'egida europea, mentre in Libano l'egida è della NATO. Anche questa è una piccola inesattezza che un Presidente del Consiglio dovrebbe evitare di commettere. Ma il discorso

che mai troverà l'accordo e avoca a sé il diritto di prendere la decisione, il che è veramente ridicolo. Nel campo della difesa e della sicurezza i prossimi nodi saranno l'Afghanistan e altri temi del genere. Come pensate di superare il problema di tutti coloro che ancora oggi dichiarano, *apertis* *verbis*, che non sono assolutamente d'accordo nel sostenere le operazioni in Afghanistan? Come pensate di far cambiare idea a coloro che vi aspettano al varco perché approvarono la volta precedente il finanziamento della missione in Afghanistan, ma in quanto avevate promesso loro una *exit* *strategy* in questo decreto? Come pensate di tacitare coloro che hanno sfilato in testa al pittoresco corteo di Vicenza, che ben poco aveva a che vedere con la maggioranza della popolazione di quella e che hanno sventolato bandiere antigovernative, offeso anche lei, signor Presidente del Consiglio, offeso il Governo, offeso gli Stati Uniti, dichiarato di voler andare via dall'Afghanistan? Come pensate di cambiare l'atteggiamento di tutte queste persone e di non riproporre la stessa situazione che si è proposta in occasione delle due risoluzioni bocciate?

quindi, un problema di coalizione, esiste un problema di individualità che rispondono a certe frange della sua compagine governativa che, come diceva bene il senatore Malan, o sono tradite o sono imbrogliate. Non c'è assolutamente dubbio.

Francamente, è veramente durissimo, è veramente difficile. Perché allora, a un certo punto, non prendere atto della realtà e ridare la voce al popolo, cioè a chi detiene il potere? a chi detiene il potere? La legge elettorale è una legge che va bene come le precedenti. Siamo l'unico popolo che ha cambiato tre leggi in poco tempo e non gliene va bene nessuna: la Germania non l'ha cambiata, la Francia non l'ha cambiata, gli Stati Uniti non l'hanno cambiata. Non solo, alcuni di noi vogliono un sistema alla tedesca, altri alla francese. Ma facciamola finita una buona volta! D'altra parte, anche le leggi degli altri Paesi creano delle situazioni di contrasto proprio in sé. Il Presidente degli Stati Uniti ha la minoranza del suo partito nel Congresso. Quante volte la Francia ha avuto il Presidente della Repubblica che non aveva la maggioranza nel Parlamento? La Germania ha dovuto fare un Governo di coalizione perché non vi era una chiara divisione. Italia a un certo punto si è creata questa situazione. È una situazione che mi pare francamente insostenibile perché, se foste veramente compatti, potreste anche tirare avanti. Allora ritorniamo alle elezioni. D'altra parte, signor Presidente del Consiglio, mi ascolti un attimo: è veramente strano che, nel momento in cui lei elenca i punti salienti del suo programma e parla, assieme a coloro che la sostengono, di un grande slancio di ripartenza e di una gran voglia di portare a termine i programmi, concluda il suo discorso dicendo che, però, il punto numero uno, il punto fondamentale, è rappresentato dal cambiamento della legge elettorale. Ma, scusate, quale Presidente del Consiglio o quale Governo, nel momento in cui dice di ripartire per dare slancio alla sua azione ed elenca i punti programmatici, pressoché all'inizio della sua legislatura, viene a raccontare che il primo punto è il cambiamento della legge elettorale che lo ha fatto eleggere? Allora, evidentemente, anche nel suo intimo sa che deve andare presto alle elezioni, probabilmente non le va di andarci con questa legge (che tra l'altro, come ha ricordato Malan, contiene tutti i punti che lei ha indicato come punti da raggiungere) e allora sostiene che il primo punto del suo Governo, dopo tutto quello che ci ha detto, è quello di cambiare la legge elettorale. Francamente, è la prima volta che mi è dato di sentirlo in un discorso di un Presidente del Consiglio che parla del programma a venire. Penso quindi che la cosa migliore sia quella di finirla con questo atteggiamento preagonico, che dà soltanto grande tristezza a tutti i nostri cittadini. Con senso di responsabilità e di *fair play* play* ridiamo il potere al popolo e il popolo si esprima, e forse questa volta si esprimerà un po' meglio.

signor Presidente del Consiglio, la sua presenza in Senato avviene dopo due clamorose sconfitte sulla politica estera subite prima dal Ministro della difesa e, subito dopo, dal ministro degli affari esteri D'Alema. Prima dell'epilogo di questa vicenda il ministro D'Alema aveva solennemente affermato che se un Governo non ha una maggioranza sulla politica estera è bene che vada a casa. Lei con le dimissioni ha fatto semplicemente finta di andare a casa. Oggi si presenta al Senato per chiedere la fiducia, una fiducia che è probabile che lei ottenga, ma che già si preannuncia solo numerica, non politica. Intatte rimangono, infatti, le riserve giù espresse da alcuni senatori della sinistra e nuove sono le riserve di alcuni senatori a vita, i quali finalmente hanno preso coscienza che una maggioranza parlamentare che si fonda sul loro voto determinante pone un problema politico non superabile. Tradotto in termini più chiari: anche se il suo Governo ottiene la fiducia sul piano numerico, se ne deve comunque andare a casa se il voto dei senatori a vita è determinante. Ora, noi capiamo la sua posizione, quella della disperazione che di fronte al fallimento della sua azione politica tenta in tutti modi di galleggiare, pur nella consapevolezza di essere a capo di un Governo, ammesso che questo Governo si possa considerare tale, paralizzato per le forti divisioni sulle grandi scelte di politica estera e di politica interna. Quello che rimane un fatto assolutamente inconcepibile è la posizione assunta dal ministro D'Alema, che, smentendo quanto ha detto una settimana fa, si presta alla riesumazione di un Governo che non c'è. Un Governo che non c'è perché la reiterazione delle posizioni espresse da alcuni senatori della sinistra conferma ancora oggi la mancanza di una maggioranza sulla politica internazionale. Non credo si possa sostenere che oggi il quadro è mutato perché un transfuga si appresta a mettere di mezzo l'Italia e gli italiani. In realtà, anche questo transfuga con la sua astensione della settimana scorsa non ha assolutamente condiviso le linee di politica estera del suo Governo. D'Alema è persona troppo seria per non capire che siamo di fronte a una grande commedia, dove il "teniamo famiglia" prevale sulle regole democratiche e sui reali interessi del Paese. Una commedia dove i Ministri dicono una cosa e poi ne fanno un'altra, una commedia dove si manifestano capriole e comprimari voltagabbana, dove il Presidente del Consiglio, con grande cinismo, continua a fare il direttore di un'orchestra cui i musicanti se la suonano e se la cantano a proprio piacimento, portando il Paese allo sfascio e facendo ricorso alla canna d'ossigeno dei pendolari della politica. Questa è la realtà, caro Presidente. Un sussulto di dignità avrebbe dovuto imporre di mantenere le dimissioni e non di mettere in atto una farsa penosa per lei, signor Presidente, ma soprattutto per il Paese. Lei, essendo un Presidente senza partito, nella consapevolezza che la sua uscita di scena sarà definitiva, allunga inutilmente la sua agonia, giocando sulle paure, sulle profonde debolezze dei suoi alleati e sul ricatto politico del «Tutti a casa» o del «Dopo di me il diluvio», con una supponenza e un'arroganza insopportabili anche per i suoi alleati, dietro le quali si nascondono idee e programmi tanto nebulosi quanto estremamente dannosi, come dimostra il suo evanescente decalogo. Andrea Romano, nel suo libro «Compagni di scuola», ci ricorda che c'è in Italia una generazione politica che ha attraversato l'ultimo ventennio, volendosi mostrare sempre unita e coesa a dispetto dei conflitti interni da cui è stata lacerata e dalle trasformazioni che hanno mutato il volto del Paese. Romano aggiunge: «È la generazione dei post-comunisti, l'ultimo gruppo dirigente del PCI e l'unica *leadership* che abbia guidato fino ad oggi i Democratici di sinistra. Una famiglia, più che una classe politica, impegnata a tutelare se stessa e la propria identità dalle minacce esterne e dalla sfida del cambiamento che, venti anni dopo la fine del PCI,» - aggiunge sempre Romano - «si avvia a concludere mestamente senza lasciare un'eredità davvero vitale». Non posso credere che il ministro D'Alema rinunci a trasformare una famiglia in una classe politica e voglia concludere mestamente la vicenda politica sua e del suo partito senza accogliere la sfida del cambiamento. Noi le chiediamo se di fronte all'esigenza di metter in campo politiche innovative più avanzate debba prevalere l'esigenza di governare comunque come lei sta facendo. Si deve continuare a governare condizionati dalle coincidenze aeree, dal decorso delle malattie influenzali, dall'apporto determinante dei voltagabbana e dei saltimbanchi o si deve scegliere la via per la costituzione di un quadro politico che dia stabilità e governabilità al Paese nella chiarezza e nella fermezza delle scelte? Dobbiamo privilegiare la gestione cinica del potere, abbassare la bandiera delle idee, alzare il vessillo degli opportunismi e dei tatticismi o piuttosto ritrovare il senso dello Stato e restituire nobiltà all'impegno politico? Il Governo che oggi si presenta al Senato, purtroppo, è il risultato di un calcolo cinico e per nulla ambizioso; manifesta un disegno che punta a guadagnare tempo per consentire di fare campagna acquisti, per corrompere le coscienze di chi sta dall'altra parte, per condizionare le scelte individuali con il favorire carriere negli organi dello Stato, per soddisfare vanità e sete di potere. Allora, rivolgendoci sempre a D'Alema, gli chiediamo: c'è tensione morale, c'è tensione morale, c'è tensione ideale in questa politica del Presidente del Consiglio? C'è tensione morale nello scontro, anche fisico, con chi dissente? C'è tensione morale nell'abbandono delle grandi linee di politica internazionale? C'è tensione morale nel blocco delle grandi opere infrastrutturali, nel negare una seria riforma previdenziale, nel negare una seria politica per la famiglia, nel negare una maggiore equità fiscale? C'è rigore morale nel mantenere sulle spalle dei cittadini una struttura pubblica e burocratica? pubblica e burocratica? Per impedire che la vostra parabola politica volga mestamente alla fine occorre uno scatto ideale; occorre raccogliere la sfida della nuova società, che non è più comprimibile in vecchi schemi, in categorie ormai obsolete, in vecchi riti; occorre guardare avanti con occhi e menti che, partendo dalle migliori esperienze del passato, sappiano interpretare i nuovi processi, assimilare le ansie e i desideri delle nuove generazioni per favorire la nascita e la crescita di una nuova società,

il presidente Prodi ha ribadito nella comunicazione di quest'oggi, aveva inserito nel programma dell'Unione e ha riconfermato nei cosiddetti 12 punti irrinunciabili. Mi riferisco alle reti TEN, alla tratta ad alta velocità Lione-Torino-Trieste, alla Berlino-Napoli-Palermo e, per la verità, signor Presidente, devo anche ricordarle che c'è la Genova-Rotterdam, che lei probabilmente ha dimenticato, ma che rappresenta una delle priorità inserite dall'Unione Europea. Con quello che sta accadendo nel mondo, con l'esplosione dei traffici marittimi, con l'affermazione della Cina, con ciò che sta diventando il canale di Suez, ignorare il potenziale di crescita dei porti del Nord, signor Presidente, oltre che di quelli del Sud, e quindi la posizione strategica di Genova e dei porti liguri, a me pare di per di per sé un peccato grave. Lei ha ribadito l'impegno politico a fare l'alta velocità, le reti TEN, peccato che questo impegno, signor Presidente, né da lei, né dai suo colleghi Ministri, sia stato esercitato con la necessaria coerenza;

con un provvedimento recente, pochi giorni fa, ha disposto la revoca delle concessioni proprio sulla tratta Genova-Milano e sulla tratta Milano-Verona, motivando la decisione con la necessità di fare gare europee risparmiando cospicue risorse. Il ministro Di Pietro si è avventurato in affermazioni quali «cancelliamo le opere che non sono partite», purtroppo per lui, per quanto riguarda la Genova-Milano-Novara-Rotterdam, signor Presidente, sono già stati spesi 250 milioni di euro; le Regioni Lombardia, Liguria e Piemonte hanno già approvato in Conferenza di servizi l'intero progetto; ci sono tutte le approvazioni; in finanziaria c'è da due anni uno stanziamento cospicuo. questo il ministro Di Pietro lo modifica e lo ignora. Le ricordo ancora che finora i suoi Ministri si sono distinti più che per costruire cose positive, per azioni finalizzate a cancellare il lavoro fatto dal precedente Governo: non una decisione in positivo, non un completamento di opere avviate, non un elenco diverso di priorità concordate con la Regione. Non avete, signor Presidente, con nessuna Regione del nostro Paese, concordato nuovi elenchi delle cosiddette priorità decise nel 2001, da voi tanto criticate. È vero: siete andati in giro per l'Italia - in questo Di Pietro è stato il vero *leader*, lo statista che ha illuminato il Paese - a dire che Berlusconi ha illuso gli italiani. Peccato che il Governo Berlusconi, signor Presidente, lo dico non per fare propaganda, ma per citare una cifra,

purtroppo, in questi nove mesi di investimenti non ne abbiamo visti, anzi forse a lei sarà sfuggito, ma gli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici risulta siano paralizzati. In questo quadro, si inserisce il documento-denuncia

il fatto cioè che nel 1967 sono transitate 19 milioni di tonnellate lungo l'arco alpino, nel 2002 ben 135 milioni, e soprattutto il dato di previsione che nel 2027 gli archi alpini saranno saturati dai flussi di traffico.

che, nella ristrettezza di risorse finanziarie di cui dispone oggi l'Unione Europea, i cofinanziamenti già decisi saranno confermati nei confronti di quei Paesi che, entro quest'anno, confermeranno concretamente tre condizioni per le opere previste nei progetti prioritari, e cioè l'accordo internazionale (che ci sarà), ci sarà), il piano finanziario che dimostra l'impegno dello Stato a coprire la quota non finanziata ed il consenso del territorio. Mi dice come farà a garantire queste tre condizioni, signor Presidente, con quei Ministri scellerati che con legge revocano contratti esistenti, con questo tira e molla sul territorio? Come farete a garantire ciò? Allora, dovreste essere più onesti nei confronti dell'opinione pubblica e dire che non ce la farete ad assorbire il cofinanziamento dell'Unione Europea e che rinuncerete a queste tratte. a queste tratte. Se è vero, com'è vero, che queste sono opere infrastrutturali strategiche, la strada da percorrere è un'altra, signor Presidente, e se lei la percorrerà con più decisione, probabilmente, in quest'Aula l'esistenza di una maggioranza diversa da quell'esercito di parlamentari che, nel passato, si sono sempre distinti per negare l'infrastrutturazione del nostro Paese. finestra") *(RC-SE)*. Signor Presidente del Consiglio, ho apprezzato la sua relazione, in primo luogo, per il rimando all'intreccio tra il metodo, le pratiche e i contenuti, e anche per il rilancio fermo delle aspettative che erano state riposte nell'Unione. Donne e uomini, italiani e stranieri, che vivono e lavorano nel nostro Paese e sono protagonisti di pratiche diffuse di relazione, di reciprocità tra soggetti molteplici e plurali, aspettano la nostra risposta, ci guardano e ci ascoltano. Nei loro confronti serve continuità di relazione e di ascolto. Si aspettavano e si aspettano un cambiamento della politica che è già oggi per loro e tra loro pratica concreta; si aspettano e praticano un'idea di sviluppo basata su consumi commisurati ai bisogni. Si aspettano e si impegnano per dare certezze alle giovani e ai giovani che desiderano un presente e la possibilità di progettare il loro futuro, che vorrebbero vivere una vita loro, non essere assistiti dai genitori, non doversi raccomandare, non dover chiedere favori per avere un lavoro stabile e tutelato. Si aspettano e portano avanti pratiche quotidiane di vita, perché alle donne non si continui a chiedere di supplire alle carenze storiche e strutturali del *welfare* e di sostenere, con il loro impegno e il loro voto, sistemi elettorali incapaci di assicurare anche solo una presenza equilibrata di donne e di uomini nelle istituzioni: è questione di democrazia elementare, ma è anche questione di una politica e di una cittadinanza non parziali e non dimidiate. Si aspettano, perché lo soffrono nell'esperienza quotidiana, che non si continuino a chiedere sacrifici ai lavoratori e alle lavoratrici, a pensionate e pensionati che contribuiscono, ed hanno contribuito, a costruire il benessere nel nostro Paese. Si aspettano e praticano relazioni di reciprocità e di mutuo aiuto, culture politiche che riconoscono e solidarizzano con l'altro da sé; tessono e ritessono legami sociali, per tenere insieme nella vita di tutti i giorni diritti sociali e diritti della persona. Signor Presidente, la maggioranza che si appresta a rinnovarle la fiducia ha il compito di incarnare un'idea di politica capace di cogliere, nella partecipazione nei corpi sociali intermedi, il volano del programma che lei ha rilanciato, fondato sulla pace, sulla non violenza, sulla libertà delle donne, sulla cooperazione e non sulla competizione che non tiene conto delle diverse collocazioni sociali. Viviamo da tempo una profonda crisi della politica istituzionale, del suo rapporto con la società, e non è solo questione di legge elettorale, ma di rilancio del profilo politico e programmatico della maggioranza. Per questo, il rinnovo della fiducia al Governo non è per noi necessità, ma opportunità, perché la politica torni a intercettarela voglia, le pratiche, la tensione al cambiamento che attraversano il nostro Paese.